Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, come anticipato dal Presidente della nostra Assemblea, l'interpellanza riguarda l'applicazione dei benefici

per l'istituzione di un Fondo nazionale per la bonifica dell'amianto dai siti, secondo un progetto già regolato da leggi, ma

Sono stati 607.700 i lavoratori esposti all'amianto che, in base alla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale del 27

lavoratori che non hanno ancora ricevuto risposta dall'INAIL, mentre circa 116.000 domande, respinte in quanto considerate incomplete, riguardano lavoratori ex esposti all'amianto dipendenti da aziende che hanno cessato l'attività

per ottenere quanto previsto in loro diritto sulla base della legge sopra citata. Numerose sono state le sentenze a tutti i livelli, incluse quelle della Corte di cassazione, della Corte dei conti e della Corte costituzionale riconosciuto il diritto ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i pensionati *post* 1992, ad ottenere i benefìci previdenziali previsti dalla legge in oggetto. Nella maggior parte del Paese sia l'INPDAP che l'INPS, dopo le sentenze, invece di provvedere all'erogazione dei benefici previdenziali, hanno presentato ricorso in appello. Questa

avveniva sulla base di esplicito invito da parte del Governo (in questo caso, si trattava del Governo precedente). Ad oggi, anche in relazione alla recente adesione da parte degli enti di cui sopra, non sembra secondo noi, un'esplicita volontà di risolvere positivamente le controversie esistenti. Voglio ricordare unicamente che si tratta di diritti che attengono all'integrità psicofisica dei lavoratori, verso i quali dovrebbe esserci, da parte del Governo e degli organi di indirizzo, una sensibilità

lavoro, per bocca anche del Ministro, fa rispetto alle questioni della tutela della salute, della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, che rischiano di essere interpretate come buone intenzioni, ma - come si dice - di buone intenzioni sono lastricate le vie dell'inferno.

se la situazione corrisponde a quanto a noi risulta e, in caso affermativo, quali sono le iniziative che avete assunto o intendete assumere, per quanto di vostra competenza, per risolvere tali problemi.

e quali misure abbia adottato affinché gli Uffici provinciali del lavoro provvedano a fornire la documentazione sui rapporti di lavoro per gli ex dipendenti delle aziende che hanno cessato l'attività; se ritenga giusto, alla luce delle varie sentenze emesse dalla Corte dei conti, dalla Corte di cassazione, dalla Corte costituzionale,

invitare gli enti previdenziali in questione a erogare le prestazioni, come definito dalle sentenze di primo grado,

il Ministero intenda adottare per favorire il rapido esame ed evasione delle domande da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, nonché l'erogazione delle prestazioni da parte degli enti previdenziali competenti, in modo da favorire la rapida soluzione dei casi controversi. non ritenga opportuno, anche alla luce delle iniziative parlamentari in atto, quanto meno sanare quegli atti di indirizzo

l'applicazione delle norme della legge in questione spesso, in alcune realtà produttive, ha comportato vere e proprie disparità

il personale, sono stati inseriti nell'elenco dei beneficiari lavoratori poco esposti, mentre altri, che lo erano stato a lungo, non hanno potuto godere di quel beneficio. Per questo riteniamo che, quantomeno nei casi più controversi, sarebbe opportuna

ne conosce la particolare rilevanza e delicatezza e per questo si è sempre dimostrato, fin dal suo insediamento, pronto ad adottare ogni iniziativa utile e necessaria a tutelare la salute dei lavoratori esposti all'amianto e a garantire la la possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge. È una vicenda complessa quella dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto e la normativa non sempre ha aiutato a garantirne i diritti. Ci sono stati

Sul piano normativo, il decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 (di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003) ha operato un sistematico coordinamento tra lo stesso articolo 47 e l'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003 e rappresenta, quindi, il quadro di riferimento normativo in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Per quanto riguarda le procedure di accertamento e di certificazione dell'esposizione all'amianto, il decreto stabilisce che «continuano a trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina: il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e documenti ritenuti utili dall'Istituto stesso. L'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicabili nell'azienda stessa». Secondo l'Istituto, il dato - menzionato nell'interpellanza - di 607.000 domande di benefici previdenziali presentate da lavoratori ex esposti all'amianto dall'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 risale a rilevazioni effettuate in una fase immediatamente successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse (15 giugno 2005), sulla base di conteggi manuali della documentazione pervenuta, effettuata dalle Unità territoriali. In seguito, le Sedi hanno inserito le nuove domande nella procedura informatica: a febbraio 2007, le domande complessivamente in carico all'INAIL - evase e non - erano 542.100, decurtate delle 30.700 trasferite per competenza all'IPSEMA (legge finanziaria 2006) e delle domande doppie presentate presso più Sedi. L'INAIL ha precisato che le certificazioni fino ad ora rilasciate - sia positive, sia negative - fanno riferimento a periodi lavorativi e non alle domande; di ciò si deve tenere conto, in quanto una domanda può generare diverse certificazioni, nei casi in cui il lavoratore abbia svolto attività presso diverse aziende. Per quanto concerne il rilascio dei *curricula* da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile (come previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 27 ottobre 2004), si fa presente che le Direzioni provinciali stanno evadendo le richieste dei lavoratori. Lo stanno facendo, però, con enorme ritardo rispetto alla data in cui le domande sono state presentate; inoltre sottolineare che un'attivazione particolare - come riferirò in seguito - si è verificata dal momento in cui si è insediato il Governo Prodi. infatti, in alcune sedi, ha avviato tavoli di confronto tra i vari organismi pubblici interessati, al fine di facilitare la sinergia tra i diversi ruoli dei soggetti tenuti agli adempimenti di legge, conseguendo considerevoli risultati positivi per la definizione delle pratiche. Relativamente, invece, alle pratiche rimaste ancora inevase, il Ministero intende continuare ad attuare il controllo e la vigilanza nelle sedi ove permangono problemi irrisolti, anche attraverso una concertazione a livello nazionale con l'INAIL e con gli altri organismi pubblici interessati alla vicenda. In merito alla rappresentata opportunità di interventi di sanatoria sugli atti d'indirizzo a suo tempo emanati, si fa presente che detta prassi è stata superata dall'articolo 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002, che ha cristallizzato l'azione amministrativa in precedenza assunta in materia, munendola, peraltro, di relativa copertura finanziaria (articolo 39, comma 3, della Relativamente ai ricorsi in appello da parte dell'INPS e dell'INPDAP, si ribadisce l'intenzione del Ministero di non invadere la sfera di autonomia gestionale degli enti previdenziali, anche in considerazione della responsabilità che grava sui responsabili dei medesimi e che potrebbe nascere dalle scelte relative alla condotta processuale da tenere con riferimento a singole vicende giudiziarie. Peraltro, proprio in ragione della ricordata rilevanza della problematica, il Ministero ha comunque intenzione di interpellare gli istituti previdenziali competenti ed acquisire ogni utile elemento di valutazione, al fine di monitorare l'evoluzione della questione, così da ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela della salute dei lavoratori ed il dovuto rispetto alla sfera di autonomia dei predetti enti. A conclusione della risposta all'interpellanza, che pone problemi molto delicati e molto complessi, devo dire che nei tavoli che sono stati attivati si è costituita una sorta di *task* *force* tra i diversi soggetti istituzionali che non avevano condiviso le responsabilità previste dalla normativa, soprattutto per quanto riguarda le aziende cessate, fallite o irreperibili, i cui lavoratori erano impossibilitati ad avere il *curriculum* lavorativo e quindi ad avere una risposta da parte delle istituzioni. Sono stati attivati tavoli in Sicilia, nelle sedi in cui maggiormente questo problema è stato sottolineato e segnalato, ma si sono aperti anche tavoli in altre Regioni del nostro Paese proprio perché riteniamo che sia indifferibile ed ineludibile la responsabilità delle istituzioni di garantire una risposta alla domanda che pongono i lavoratori. Su questo aspetto assicuro il senatore Tibaldi che sarà fatto un monitoraggio su tutto il territorio nazionale, non soltanto con intese che dovranno essere fatte tra la direzione del Ministero (per quanto riguarda l'attività ispettiva e l'INAIL e, per quanto riguarda l'IPSEMA, anche l'IPSEMA), ma anche in sede territoriale, in modo da mettere in coordinamento le attività dell'INAIL con le Direzioni provinciali del lavoro per garantire al più presto che tutti i lavoratori possano avere la risposta più adeguata rispetto al loro diritto.

mi ritengo parzialmente soddisfatto soprattutto per la volontà manifestata dal Ministro

mi preme sottolineare che è vero che i dati citati sono risultati inferiori, che probabilmente le lavoratrici e i lavoratori interessati saranno ancora

in modo che si riesca, laddove le aziende non esistono più, a fornire una certificazione sufficiente utilizzando anche le testimonianze dei lavoratori; cose che tutti conosciamo. Mi lascia un po' un po' perplesso la sua affermazione riguardante l'autonomia dei singoli enti: ogni ente è autonomo e il Ministero non può decidere cosa deve fare in termini di ricorsi. In questo In questo caso, però, voglio ricordarle che, per dichiarazioni rilasciate dai massimi responsabili degli enti, la pratica di tirare in lungo il mancato riconoscimento, e quindi di fare ricorso, era adottata su precisa indicazione del Ministero del tesoro del Governo precedente.

Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione in discussione, relativa alla società Cucirini Cantoni Coats, dalle notizie fornite dal Dipartimento Servizi ai cittadini-Servizio lavoro della Provincia di Lucca e dagli accertamenti esperiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Lucca è emerso quanto segue. L'azienda in questione, appartenente al Gruppo Coats Cucirini Srl, con sede legale in Milano, attualmente di proprietà estera, con sede operativa in Lucca presso gli stabilimenti della località Acquacalda, concentra storicamente nel territorio della Provincia il più importante complesso produttivo del settore tessile per la fabbricazione di filati. Negli anni a seguire, Settanta e Ottanta, a causa dei processi di ristrutturazione del settore manifatturiero generale e in particolare del tessile si è assistito ad un progressivo taglio delle produzioni e dei livelli occupazionali che di fatto hanno sempre più diminuito l'interesse industriale per la nota fabbrica di Lucca. Negli ultimi anni c'è stato un progressivo spostamento di alcune produzioni e talora di intere filiere verso Paesi orientali dove, è risaputo, il costo della manodopera, anche se non sempre specializzata, è notoriamente più basso. La proprietà attuale del gruppo Cucirini Cantoni ha deciso nel corso di questo inizio del 2007 e nel quadro di un progetto di un globale riassetto produttivo che ha coinvolto anche altri stabilimenti presenti in Italia, di procedere progressivamente ad una chiusura delle linee produttive di Lucca per lasciare solo le attività relative alla gestione del magazzino dei prodotti filati domestici. I primi segnali di grave preoccupazione sul futuro dell'attività produttiva si erano avvertiti a partire dal dicembre del 2006 quando la proprietà ha deciso di vendere lo stabilimento dell'Acquacalda ad imprenditori lucchesi, rimanendo l'azienda in rapporto di locazione degli immobili per due anni. Il Consiglio provinciale di Lucca, nella seduta del 26 febbraio 2007, aveva espresso all'unanimità il sostegno ai lavoratori e alle lavoratrici ed aveva impegnato la Giunta provinciale ad intraprendere con il Comune di Lucca e la Regione Toscana tutte le iniziative necessarie per il mantenimento dell'attività manifatturiera tessile e la difesa dei posti di lavoro. Successivamente, nei primi giorni di marzo 2007, la proprietà ha annunciato l'avvio delle procedure di mobilità per 140 dipendenti, per la metà con età inferiore a trentacinque anni, e con una presenza femminile pari a 86 unità. Voglio sottolineare che questa è un'azienda che vede una massiccia presenza femminile. Immediatamente le organizzazioni sindacali hanno indetto una manifestazione di sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della Cucirini e di protesta per gli annunciati licenziamenti, che si è svolta il giorno 7 marzo 2007 presso la sede di Palazzo Ducale della Provincia di Lucca, in occasione di un incontro appositamente convocato per fare il punto sull'annunciata crisi occupazionale e sulle iniziative di natura istituzionale da intraprendere. In questa sede si è convenuto di avviare l'apertura di un tavolo istituzionale che coinvolgesse parti sociali, istituzioni e lavoratori al fine di scongiurare la dismissione dello stabilimento e garantire al massimo livello tutte le tutele di garanzia previste per la salvaguardia dei diritti degli stessi lavoratori. Contestualmente, si è deciso dì convocare la proprietà del gruppo Cucirini Cantoni Coats in un incontro, fissato per il giorno 12 marzo 2007 presso la Regione Toscana. Durante la riunione è emersa la volontà, da parte della proprietà, di confermare la chiusura dello stabilimento per le attività produttive, stante la non competitività dei costi di produzione - queste le ragioni addotte dall'azienda - ed il calo delle vendite della produzione di Lucca, e di lasciare quindi soltanto le attività del magazzino, limitatamente ai prodotti domestici, per un impegno di circa 50 dipendenti. Si è tuttavia riscontrata un'apertura, da parte del gruppo Cucirini, ad avviare un percorso di ammortizzatori sociali più consono alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici, che prevedesse anche la cassa integrazione straordinaria per favorire il pensionamento di un certo numero di unità di lavoratori. A seguito di questa riunione, sono iniziate le trattative (durate circa 25 giorni) fra azienda e sindacati, con l'intervento dell'Associazione industriali, per definire il contenuto di un accordo sindacale,

Tale accordo prevede il licenziamento di 89 unità a partire da luglio 2007, in maniera graduale e con il ricorso, oltre che alla mobilità incentivata, anche alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione parziale di attività, ai sensi del decreto ministeriale 31826 del 18 dicembre 2002, onde consentire la maturazione dei requisiti di pensionamento o la ricerca di una ricollocazione lavorativa. La collocazione in CIGS avverrà gradualmente entro il mese di luglio prossimo venturo, in relazione alla graduale cessazione dell'attività produttiva ed al conseguente smantellamento delle attrezzature per il loro trasferimento altrove e dopo che i dipendenti interessati avranno fruito delle ferie e dei permessi retribuiti loro spettanti. I lavoratori che rimarranno nell'azienda saranno impiegati nell'attività del magazzino, per il quale l'azienda si è impegnata ad una nuova localizzazione per un'area di circa 7.000 metri quadrati, da realizzare entro l'agosto del 2008 nel territorio provinciale, continuando ad operare negli attuali locali fino alla realizzazione del predetto trasferimento. Inoltre l'azienda si è impegnata, nei mesi di maggior lavoro, a riassorbire i lavoratori messi in mobilità per consentire loro la maturazione di ulteriori periodi di pensionamento.

ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori che fuoriescono dall'azienda e, dall'altro, insieme al Ministero per lo sviluppo economico, per verificare se e quali spazi ulteriori ci sono. Naturalmente

Non è casuale che il più grande produttore della materia prima, cioè il cotone, di cui il Brasile e i Paesi africani hanno denunciato un'infrazione commerciale, siano gli Stati Uniti d'America: una qualche ragione c'è.

un pezzo della loro produzione, della loro industria, della loro capacità di intervenire sulle materie prime insieme al rapporto con i Paesi in via di sviluppo.

le varie istituzioni locali, perché immagino che il prossimo passo sarà il cambio di destinazione d'uso dei vecchi capannoni e la costruzione di centri commerciali. È curioso sapere che in

lei come me, è assolutamente conscio che lo svolgimento nella seduta di oggi dell'interpellanza urgente presentata da 40 nostri colleghi senatori avrebbe buoni motivi per essere considerata superflua. Nell'atto di sindacato ispettivo si domandavano al Governo chiarimenti sul mancato invio al Parlamento del rapporto sulle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti che, a norma di legge, l'ARAN deve trasmettere al Parlamento ogni tre mesi e, soprattutto, si chiedeva al Governo se riteneva opportuno, «definire la propria strategia negoziale nell'imminente stagione di rinnovo dei contratti pubblici anche alla luce dei dati relativi all'andamento delle retribuzioni di fatto dei dipendenti pubblici negli ultimi anni». Con la stipula Con la stipula alla vigilia di Pasqua, al riparo dall'attenzione dell'opinione pubblica, dell'ennesimo protocollo d'intesa con i sindacati del pubblico impiego il Governo ha evidentemente risposto: no, l'Esecutivo non ritiene che i dati sugli aumenti effettivamente percepiti dai pubblici dipendenti negli ultimi anni debbano essere tenuti in considerazione in sede di definizione contrattuale. O forse, più probabilmente, il Governo ben conosce i dati e, proprio perché li conosce, ritiene opportuno che non vengano resi pubblici e ufficiali. nonostante l'atteggiamento farisaico del Governo, il tema sollevato resta quanto mai attuale e diventa, anzi, ancora più urgente alla luce dell'avvenuta stipula dell'intesa tra Governo e sindacati. Il tema delle risorse da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego non solo è rilevante in termini di equilibrio della finanza pubblica, ma soprattutto è una questione di equità sociale che il Governo di centro-sinistra, questo Governo, si rifiuta di garantire. Non è uno *slogan*, ma una tesi supportata da dati e prove inconfutabili. Nel periodo 2000-2005, infatti, le retribuzioni di fatto del settore pubblico sono aumentate quasi del 24 con punte del 25,8 nelle amministrazioni centrali e del 26,8 negli enti locali: il triplo rispetto all'inflazione programmata dell'8,4, il doppio dell'inflazione effettiva del 12,6 e quasi il doppio delle retribuzioni del settore industriale nelle quali l'aumento è fermo al 15,1. I dati diventano ancora più drammaticamente eloquenti se consideriamo, come il rapporto ARAN del quale siamo vanamente in attesa dovrebbe correttamente fare, anche i dati del 2006. Considerando che l'anno scorso sono andati in esecuzione praticamente tutti i contratti collettivi relativi al biennio 2004-2005 con aumenti medi del 5,01 per cento, l'aumento complessivo del periodo 2000-2006 è stato superiore al 30 il doppio rispetto ai salari del settore privato. Se questi dati non pongono un problema di equità tra chi il lavoro stenta a trovarlo, tra chi il lavoro ce l'ha ma deve ogni giorno augurarsi che l'azienda per cui opera non lo licenzi o lo metta in cassa integrazione, integrazione, se non addirittura fallisca e chi invece, dipendente della pubblica amministrazione, è consapevole di appartenere ad una categoria protetta, a rischio quasi zero di licenziamento dove il cattivo esempio di pochi fannulloni invita i propri colleghi ad un dolce far niente, anziché spronarli a dimostrare di essere più capaci, non so quale altro esempio potrebbe essere più eloquente. Non si tratta solamente di un pessimo esempio di cattiva allocazione delle risorse, ma la prova tangibile che questo Governo è sotto il ricatto del sindacato del pubblico impiego. L'incapacità di essere reale e capace controparte negoziale nelle trattative è anche confermata dalla pantomima del conflitto minacciato dai rappresentanti dei lavoratori pubblici. Perché, nei fatti, il sindacato ha chiesto ciò che sapeva avrebbe ottenuto e il Governo è stato impossibilitato a dire di no, per evidenti ragioni di equilibrio politico o anche solo a pretendere, come contropartita, un confronto serio sulle inefficienze economiche e funzionali della nostra amministrazione Si è così sottoscritto l'ennesimo protocollo, questa volta sulle risorse da destinare ai rinnovi, dopo aver firmato un *memorandum*, quello di gennaio 2007, che di fatto consegnava al sindacato anche le iniziative di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che - come detta il *memorandum* - devono essere «concordate in connessione con il rinnovo dei contratti». rinnovo dei contratti». Traduciamo in italiano: si è così delegata l'organizzazione e il potere di riforma, fin qui riserva di legge, alle organizzazioni sindacali. Così come rappresenta un'ennesima concessione al sindacato che i dirigenti, già deboli, nell'adottare il piano operativo «concordino obiettivi e modalità con le parti sociali». con le parti sociali». Anche ciò, finora, non era mai avvenuto. Ovviamente restiamo in viva attesa di conoscere gli atti di indirizzo che il Governo emanerà per avviare la nuova stagione contrattuale al fine di valutare quanto delle prerogative del legislatore il sindacato avrà avocato a sé. Su questo aspetto, come spetta a una opposizione seria, annunciamo fin d'ora che daremo battaglia. Ma la vicenda di un rapporto che l'ARAN sarebbe obbligata a inviare ogni tre mesi al Governo e al Parlamento e che, invece, non viene pubblicato per evitare al Governo di giustificare al Parlamento e all'opinione pubblica i perché il pubblico impiego venga privilegiato rispetto ad altre categorie, e per evitare al sindacato la difficoltà a invocare aumenti non giustificati dalle cifre, ha una sua emblematicità. Peraltro, non è neppure vero che bisogna sempre guardare con favore risorse aggiuntive che si rendono disponibili. Se esse fossero illimitate nessuno negherebbe rinnovi contrattuali a a nessuno. Ma visto che così non è, un Governo che si rispetti dovrebbe saper soddisfare invece quei bisogni che al momento appaiono prioritari. E francamente il rinnovo dei contratti, se non per ragioni elettoralistiche, non appare affatto prioritario. E non ci sia venduta la frottola ricorrente, secondo la quale gli aumenti registrati sarebbero il frutto dei ritardi accumulati nella stipula di contratti della passata legislatura, perché i ritardi possono essere stati anche considerevoli, ma i sindacati sanno benissimo che hanno percepito fin all'ultimo euro computato alla data dell'inizio della stagione contrattuale e non alla data della stipula del nuovo contratto (circostanza che, invece, si verifica puntualmente nel settore privato). Del resto, il balletto di cifre a cui siamo abituati da tempo, in un classico gioco delle parti dove il sindacato "gioca" con i dati relativi alle retribuzioni contrattuali, facendo finta di ignorare le risorse che vengono distribuite in sede di contrattazione decentrata (la cosiddetta contrattazione integrativa), non fa altro che avvalorare la tesi per cui la condizione di "trattativa permanente" con il sindacato alla quale questo Governo ci ha abituato è funzionale ad accontentare quello che risulta essere il suo vero azionista di riferimento. Ricostruiamo brevemente le tappe di questa contrattazione permanente. Si è iniziato con la sostituzione dei vertici ARAN. Si è poi proseguito con la trattativa in sede di approvazione della legge finanziaria 2007 concedendo l'emendamento cosiddetto "salva contratti", che traduceva in legge un accordo che, oltre a garantire la stipula dei contratti anche a costo di pregiudicare la compatibilità economica degli stessi con gli obiettivi di finanza pubblica, chiariva anche che tutte le risorse stanziate dalla finanziaria erano riferibili al biennio 2006-2007 (anche la quota la cui decorrenza era fissata al 1° gennaio 2008). In sostanza, il sindacato otteneva che venisse inequivocabilmente precisato che non vi fosse lo slittamento di un anno del biennio contrattuale, e il Governo difendeva gli equilibri della manovra, dichiarando solennemente che l'accordo raggiunto non avrebbe comportato alcun onere per la finanza pubblica (si veda a proposito la relazione tecnica trasmessa dal Governo alla Commissione bilancio). Ovviamente, sappiamo che la dichiarazione era falsa. Il maggior onere per la finanza pubblica c'è ed è anche quantificabile in almeno 3,7 miliardi di euro (sarebbero 2 miliardi se considerassimo solo gli statali, ma il dato è fuorviante perché i contratti riguardano in realtà tutto il pubblico impiego). Nonostante dunque il Governo dichiari che il tesoretto del ministro Padoa-Schioppa, ottenuto grazie alla politica economica del Governo precedente, non sarà destinato ai rinnovi contrattuali, siamo ben consapevoli che imputare (solo contabilmente) le risorse necessarie al 2008 è un espediente contabile che trasla al prossimo anno, alla prossima finanziaria, un onere eccessivo per la nostra finanza pubblica. Sottrarre fin d'ora risorse al prossimo anno è un mezzuccio per destinare il tesoretto già da oggi, senza però darlo ad intendere. In quest'ottica è evidente che il monito lanciato ieri dal Fondo monetario internazionale in merito alla necessità di ridurre il debito è già diventato, oggi, lettera morta. morta. Così, la semplice minaccia di uno sciopero generale (dall'esito quantomeno incerto) a ridosso delle elezioni amministrative ha raggiunto il suo scopo. Anzi, c'è da attendersi che il sindacato non si accontenti dei soldi offerti dal ministro Nicolais, ma pretenda qualcosa in più, con buona pace del risarcimento sociale invocato da Rifondazione comunista (a meno di non ritenere che i soggetti da risarcire siano i tre milioni e mezzo di impiegati pubblici, molto protetti e assai poco usurati). In quest'ottica deve leggersi l'atteggiamento miope del Governo - e vengo alla seconda interpellanza - sulla questione da noi sollevata; esso avrebbe avuto tutto l'interesse, teorico s'intende, a sollecitare l'ARAN a divulgare per tempo (siamo già a oltre otto mesi di ritardo) il nuovo rapporto trimestrale, ma l'atteggiamento invece dimostrato fino a oggi è la conferma che, nonostante l'intuizione del 1993 di creare un agente negoziale unico che desse reale rappresentatività alla parte datoriale pubblica, l'ARAN è cosa del sindacato. Lo è da quando essa è stata istituita, tranne una breve parentesi sul finire della passata legislatura, signor Presidente, parentesi in cui, per la prima volta,

Del resto, non a caso, la prima cambiale messa all'incasso dal sindacato, all'indomani dell'insediamento del nuovo Governo, è stata, come si è detto, la sostituzione del vertice ARAN con uno più in sintonia, per usare un eufemismo, con le organizzazioni sindacali, nonostante le assicurazioni fornite a questo Parlamento in sede di Commissione dal ministro Nicolais che ciò non sarebbe avvenuto. Abbiamo infatti assistito ad una scelta del Governo, forse illegittima, visto che la legge fissa per il vertice dell'Agenzia una chiara incompatibilità con l'assunzione di incarichi sindacali, ma senz'altro inopportuna. a smentirmi, sostenere che il coordinatore editoriale della rivista culturale della CGIL «Quaderni di rassegna sindacale» non sia *embedded* (per usare un termine in voga) con il sindacato, oppure che l'ex segretario confederale per il pubblico impiego della UIL, in quanto non più in carica, possa ritenersi, oggettivamente, non in conflitto di interessi con la carica rivestita. siamo ampiamente persuasi che l'occultamento dei dati contenuti nella relazione trimestrale sull'andamento delle retribuzioni, così come l'accettazione di una situazione di egemonia del sindacato sull'agente negoziale che rappresenta la parte pubblica, siano in primo luogo dannose per il Governo. Lo sarebbero per qualunque Governo, ma lo sono a maggior ragione per un Governo di sinistra. Maggiore trasparenza dei dati, maggiore autonomia dell'ARAN avrebbero aiutato questo Governo a resistere a pressioni sindacali e ad elevare il profilo riformista della propria azione. In ogni caso si tratta di scelte che non giovano al bene pubblico, e sono contrarie a quel codice etico, minimo e condiviso, che dovrebbe guidare ogni Governo della cosa pubblica, di destra o di sinistra che sia. II Governo ha il dovere, per il rispetto che il Parlamento pretende, di operare nel modo più celere possibile affinché l'organo della sovranità statale possa essere messo nelle condizioni di valutare i dati relativi all'andamento delle retribuzioni di fatto nel pubblico impiego, avendo cura di sollecitare l'ARAN a diramare in tempi brevi l'ultimo rapporto trimestrale con la cortese, ma ferma richiesta che i dati in esso contenuti siano aggiornati e completi per ciascun comparto di contrattazione. La richiesta non è senza ragioni, poiché non vorremmo che tra qualche giorno vedessimo pubblicato un rapporto trimestrale con dati aggiornati al settembre-ottobre 2006 (dati da diverso tempo disponibili e quindi non certo i più attuali). Vorremmo invece che il rapporto ARAN contenesse un'analitica raccolta dei dati aggiornati a tutto il 2006 così che il Parlamento possa valutare compiutamente l'andamento delle retribuzioni di fatto (che sappiamo essere cosa diversa dalle retribuzioni contrattuali che non tengono conto della cosiddetta contrattazione integrativa - tanto per intenderci la contrattazione che avviene a livello decentrato presso le singole amministrazioni e che la Corte dei conti ha da tempo indicato come uno dei buchi neri della finanza pubblica, territorio in cui i sindacati «aziendali» del pubblico impiego spadroneggiano). Paradossalmente proprio oggi a pagina 2 de «Il Sole 24 ORE» leggiamo che davanti al tentativo del Governo di porre freni alla Contrattazione integrativa la levata di scudi del Sindacato ha costretto il ministro Nicolais a dichiarare che si consente «l'utilizzazione dei fondi delle singole amministrazioni nell'ambito delle proprie risorse di bilancio per conseguire ulteriori miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi». *Ergo*, niente *Ergo*, niente limiti alla Contrattazione integrativa! Il ministro Nicolais è di Napoli come me, conosce benissimo il significato dell'espressione «fuga francese, ritirata spagnola», non capisco veramente per quale motivo voglia diventarne uno specialista: è la terza o quarta volta che produce delle marce avanti per poi fare delle subitanee marce indietro. Allo stesso modo, e anche a nome dei colleghi firmatari della interpellanza urgente che oggi si discute, inviterò il Presidente del Senato a farsi garante delle prerogative costituzionali del Senato della Sarebbe importante che anche da parte sua venga sollecitato il Governo nella vigilanza dell'attività dell'ARAN e, nei confronti della stessa Agenzia, che venga rispettato il dettato normativo che prevede che il rapporto trimestrale venga inviato ai Presidenti delle due Camere per l'inoltro alle Commissioni permanenti competenti per materia. In tal senso ho già inviato un'esplicita richiesta all'onorevole presidente

toni decisamente non noiosi, evitando di assumere l'atteggiamento del mero lettore di appunti, così come notoriamente ci capita di fare, anche se è una lettura consapevole e condivisa.

di accettare l'invito da lei rivolto al Governo per il tramite della mia modesta persona, dicendole subito che, al di là del suo diritto a sfidare l'Esecutivo, non accolgo tale sfida, non perché non abbia argomenti da opporre, ma perché lo spirito con il quale assolvo a questa funzione temporanea, non è certamente quello di una contrapposizione tra nemici,

Vorrei subito chiarire, senatore Quagliariello, che non mi pare farisaico l'atteggiamento del Governo, perché

abbia potuto esprimere le sue buone ragioni di candidato al Senato, opponendole a quelle di un altro cartello politico che aveva un proprio programma. Il Governo sta attuando il programma; l'espressione «farisaico» si addice a quanti peccano di incoerenza, a quanti dichiarano di voler assumere un atteggiamento ma poi, di fatto, mettono in pratica Non abbiamo detto che avremmo messo in liquidazione la pubblica amministrazione; non abbiamo detto che avremmo chiuso le porte ai sindacati; viceversa, abbiamo detto (e lo stiamo facendo) che avremmo rilanciato la pubblica amministrazione e avremmo opposto la nostra azione alle tentazioni - peraltro, purtroppo, sempre più frequenti - di parlare alla pancia della gente, presentando agli occhi dell'opinione pubblica i pubblici dipendenti come fossero dei mantenuti.

stiamo attuando una politica di riorganizzazione, riordino e rilancio della pubblica amministrazione, ben consapevoli dei limiti e delle criticità che esistono, sfuggendo però a ogni pulsione, ad ogni tentazione di utilizzare espressioni qualunquistiche per ottenere, alla stessa stregua di qualche notista giornalistico o politico, il plauso di quanti sono sensibili ai discorsi di basso profilo. Lei afferma che il Governo sarebbe sotto il ricatto delle organizzazioni sindacali. Non so cosa lei intenda con l'espressione "ricatto", intenda riferirsi a qualcosa di istituzionalmente patologico oppure ad una valutazione politica, che naturalmente volutamente e doverosamente lascio alla sua creatività politica. Non vi è alcun ricatto. Noi partecipiamo agli incontri con i sindacati, durante i quali portiamo le nostre opinioni, difendiamo le nostre posizioni e non subiamo alcun complesso di inferiorità. di inferiorità. Non abbiamo però neanche complessi di superiorità; sappiamo che le organizzazioni sindacali assolvono ad una funzione istituzionale e siamo felici di poter svolgere il nostro lavoro di Governo attuando una concertazione che altrove, quando magari si debbono attuare o portare avanti iniziative di carattere assistenzialistico, viene invocata. Lei sostiene che il rinnovo del contratto non è prioritario. Non mi passa neanche per la testa, conoscendo la sua esperienza e avendo avuto modo di apprezzare anche in altre circostanze la sua grande preparazione, il dubbio che lei possa prescindere dal significato semantico, ontologico della parola "contratto". Il contratto non è un incidente di percorso. Il contratto è un contratto: è, cioè, un rapporto bilaterale, che per definizione deve essere onorato. Nel momento in cui il Governo scopre l'ovvietà di questa condizione, non fa altro che esercitare fino in fondo il proprio dovere. Dunque, i doveri sono priorità. Ecco perché non sono d'accordo con lei, neppure su questo tipo di valutazione. Lei afferma che la decorrenza dal 2007 sarebbe una forzatura, l'esempio di un modo strumentale utilizzato dal Governo per sottrarre, in maniera surrettizia, fondi da destinare agli statali. Non mi pare vi sia niente di surrettizio. È stato stabilito che la decorrenza è dal 2007 perché il biennio è 2006‑2007. Ho soggezione ad allargarmi in questo discorso perché non vorrei commettere l'errore - da buon sardo, spero di potermi considerarmi tale, non sono certamente aduso all'adulazione - di esercitare un'azione di piaggeria nei confronti di chi così abilmente e nobilmente presiede in questo momento la seduta, quale ha affrontato i problemi del pubblico impiego portando avanti atteggiamenti anche più avanzati rispetto a quelli dell'attuale Governo. Allora, caro senatore, come funziona? Quando il Ministro era della sua parte politica, le cose andavano bene; adesso che il Ministro non appartiene più alla sua parte, lei taccia di fariseismo il Governo, afferma che esso vuole gabellare la buona fede degli italiani utilizzando altri strumenti e sostiene che i contratti non sono priorità.

anzi, lei sa benissimo - e glielo dico volentieri, senza tono di sfida, ma unicamente per voler onorare la sua intelligenza che un gran numero di precari già sanati sono il frutto di assunzioni assolutamente legittime che sono state decise e operate nella parte finale della passata legislatura, quella di cui lei ha appena tessuto le lodi. Allora, caro senatore Quagliariello, fermo restando il suo intangibile diritto (e io sarei il primo, qualora ve ne fosse bisogno, a solennizzarlo) di esercitare la sua azione di interrogante, piuttosto che accogliere la sfida, che - le ripeto - non appartiene alla mia cultura, accolgo l'invito che lei molto opportunamente rivolge al Governo per un'azione di riordino della pubblica amministrazione. Ma noi questo lo stiamo già facendo.

forse dimentica che il precedente Presidente dell'ARAN, nobilissima persona, è stato nominato dal passato Governo, non credo né per meriti sindacali, ma neanche per meriti politici;

non lo avesse ritenuto tale, e non si può dire che in quella seduta ci fosse il governo Prodi, perché le sto parlando di una seduta del marzo 2006, quando il governo Prodi, almeno il secondo, ancora non

dell'ARAN in termini di sindacalizzazione non esiste. Infatti, al di là delle sue richieste di sfida, lei potrà verificare che all'atto dell'insediamento, o meglio della nomina delle persone che fanno parte dell'ARAN, queste non avevano in essere alcun tipo di rapporto che potesse in qualche modo inficiare la legittimità del provvedimento. Mi permetta di chiudere questo mio intervento a braccio - che lei avrà comunque la bontà di accogliere per ciò che è, vale a dire un sincero, onesto e sentito confronto sottolineando un aspetto. La penso diversamente da lei riguardo al ministro Nicolais: non gli attribuisco alcuna doppiezza, né alcuna attitudine a parlar bene e ad operare male. Non conosco la storia dei francesi e degli spagnoli di cui lei ha parlato, riferendosi alle battute che circolerebbero a Napoli, le posso però dire una cosa che riflette il comune sentire della mia terra: il ministro Nicolais non è uno che «spara da dietro i muretti a secco» e credo che questa espressione, ancorché declinata con uno *slang* diverso dal suo, sia sufficientemente chiara perché lei comprenda quanta stima io abbia del ministro Nicolais. Signor Presidente, con il suo permesso,

Come ho già avuto modo di chiarire a nome del Governo il 23 gennaio scorso, rispondendo ad un'interrogazione del senatore Sacconi su analogo oggetto, il Comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Di questi, due componenti sono designati da soggetti estranei al Governo: uno dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI, congiuntamente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia, designa gli altri tre componenti tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, il Presidente. Al momento dell'insediamento del nuovo Governo, il Comitato direttivo dell'ARAN, nominato con decreto presidenziale del 20 marzo 2006, risultava composto soltanto dai tre componenti designati dall'Esecutivo, in quanto la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e le associazioni degli enti locali non avevano indicato alcun nominativo. Peraltro, il Presidente del Comitato era stato nominato nonostante il fatto che in data 1º marzo 2006, in sede di parere della Conferenza unificata, le Regioni avessero espresso a maggioranza parere negativo e altrettanto avesse fatto, in precedenza, l'UPI - motivando lo stesso, non sulla base di un giudizio negativo nei confronti del soggetto designato, ma in considerazione delle specifiche competenze richieste dall'incarico. A ciò si aggiunga che la nomina del presidente e dei componenti del Comitato è stata effettuata ben oltre la data di scioglimento delle Camere, ovvero nel periodo sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145. Pertanto, risulta di tutta evidenza che tale assetto incompleto del Comitato non abbia potuto assicurare lo svolgimento delle attività dell'organismo stesso, in particolare nella delicata fase di avvio delle trattative relative ai rinnovi contrattuali per il quadriennio 2006-2009. Al fine, quindi, di assicurare la piena operatività dell'Agenzia attraverso la ricostituzione e integrazione del Comitato, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto del 15 novembre 2006, ha provveduto alla revoca del presidente uscente e di un componente del Comitato direttivo. Inoltre, il Comitato direttivo non era, comunque, nella possibilità di funzionare, per effetto delle dimissioni presentate dall'altro componente, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento generale di organizzazione dell'ARAN, per le riunioni del medesimo Comitato è necessaria la presenza di almeno tre componenti. Infine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2006, il Comitato è stato integralmente ricostituito, con le modalità e sulla base delle designazioni acquisite ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei requisiti professionali ivi indicati. In tale ambito, l'avvocato Massimo Massella è stato nominato presidente del Comitato direttivo, previo parere favorevole della Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato-Città, espresso all'unanimità. Per le ragioni illustrate, risulta evidente che la piena ed effettiva operatività dell'ARAN è stata ripristinata soltanto a partire dal gennaio 2007 e ciò spiega la mancata diramazione dei due rapporti trimestrali relativi al secondo semestre 2006 sull'andamento delle retribuzioni del pubblico impiego. Inoltre, si osserva che quella di diramare comunicati ufficiali da parte del Governo per dare notizia dell'avvenuta nomina dei componenti del Comitato direttivo dell'ARAN non appare essere una «prassi consolidata».

Per quanto attiene, poi, ai *curricula* del professor Mimmo Carrieri e del dottor Giancarlo Fontanelli, si tratta di esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale ed entrambi hanno all'attivo una copiosa e prestigiosa attività scientifica e professionale (il primo anche in qualità di docente universitario). A proposito del professor Carrieri, si precisa che la rivista «Quaderni di rassegna sindacale - Lavori», del cui Comitato scientifico il medesimo professore fa parte, è edita da un soggetto giuridico distinto dalla CGIL Di conseguenza, risulta che nessuno dei due suddetti componenti dell'ARAN ricopra attualmente cariche sindacali né abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni sindacali. A tale riguardo, si rammenta il contenuto dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato dall'interrogante, che al comma 7 stabilisce espressamente il divieto di essere componente del comitato direttivo dell'ARAN per coloro «che rivestano «che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni». Perché sorga l'incompatibilità a far parte del comitato occorre, quindi, che lo svolgimento di cariche o rapporti di collaborazione e consulenza con le organizzazioni sindacali sia attuale e contemporaneo alla nomina in seno al comitato. Non è invece di alcuna rilevanza giuridica il fatto di averle eventualmente rivestite in passato. Per quantoconcerne, poi, l'andamento e le dinamiche degli aumenti retributivi del lavoro dipendente, va sottolineato che esse sono identiche nel settore pubblico ed in quello privato. Infatti, l'accordo Governo-sindacati del 23 luglio 1993 prevede modalità e forme di adeguamento del salario all'inflazione reale rispetto a quella programmata identici per il settore privato ed il settore pubblico. Pertanto, in sede di rinnovi contrattuali 2002-2005, si è proceduto ai conseguenti riconoscimenti retributivi, con recupero del potere di acquisto del salario dei dipendenti pubblici nelle forme previste dal predetto accordo del luglio 1993, la cui vigenza ed effettività viene pienamente confermata anche per i prossimi rinnovi contrattuali relativi al quadriennio 2006-2009. Il Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993 è dunque lo strumento fondamentale della politica dei redditi e del lavoro sia per il settore privato che per il settore pubblico. Alla base della quantificazione delle disponibilità finanziarie per la contrattazione collettiva, individuate nelle leggi finanziarie annuali, si pone l'elaborazione del conto annuale del personale, a cura della Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta il documento contabile fondamentale ai fini della ricognizione e dell'analisi del costo del lavoro pubblico. Sulla base dei dati contenuti in tale documento avviene l'individuazione delle unità di personale in servizio e della relativa retribuzione media, in riferimento all'anno precedente a quello di inizio della tornata contrattuale. Moltiplicando i due fattori, viene definita la massa salariale esistente alla quale, in base a quanto stabilito dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993, si applica il tasso di inflazione programmato per il successivo triennio secondo le previsioni del Per quanto attiene, in particolare, alla contrattazione integrativa, si osserva che in data 11 aprile 2007 l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, presieduto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ha approvato il «Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali per il quadriennio 2006-2009», che stabilisce, tra l'altro, precisi limiti agli aumenti retributivi in sede di contrattazione decentrata. In particolare, nel documento è stabilito espressamente che l'integrazione delle risorse finanziarie per gli anni 2007 e 2008 consente di riconoscere, a decorrere dal 2008, benefici a regime nella misura complessiva del 4,46 per cento, comprensivi della quota incentivante della retribuzione, disciplinata dalla contrattazione integrativa. Nella effettiva attribuzione dei benefici economici occorrerà, inoltre, rispettare i vincoli finanziari derivanti dalle risorse attualmente disponibili. Lo stesso documento stabilisce che ai fini della destinazione di tale beneficio, e in applicazione delle regole fissate dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, nell'ambito degli atti di indirizzo settoriali dovrà essere utilizzata una quota non inferiore allo 0,5 per cento per il finanziamento dell'incentivazione della produttività e del merito secondo le indicazioni e per le finalità contenute nella "Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" del 6 aprile 2007. Gli incrementi di regime non potranno superare complessivamente il 4,46 per cento, comprensivo della quota da destinare alla produttività nell'ambito della contrattazione integrativa. Ulteriori incrementi retributivi sono espressamente esclusi dal documento che li ritiene incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica. Pertanto, la percentuale di risorse destinate ad incrementare la produttività, da individuare comunque nell'ambito del 4,46 per cento, non potrà in alcun modo essere integrata a livello nazionale né decentrato, costituendo il limite massimo, invalicabile di beneficio riconoscibile per il biennio 2006-2007. L'unica possibilità di integrare i fondi per la contrattazione integrativa è collegata al conseguimento di ulteriori *standard* di miglioramento, qualitativo e quantitativo, dei servizi pubblici erogati e comunque nel rispetto complessivo dei vincoli di finanza pubblica previsti dalle leggi e nella garanzia dell'equilibrio di bilancio. Tale limitazione, condivisa da tutti i comitati di settore partecipanti all'Organismo di coordinamento, consente per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, ivi incluso quello delle Regioni, delle autonomie locali e del Servizio sanitario nazionale, di operare politiche di contenimento dei costi del personale in base agli specifici vincoli previsti dalle recenti leggi finanziarie. Da quanto evidenziato risulta l'inesistenza di una condizione di sperequazione tra le retribuzioni dei dipendenti del settore pubblico rispetto a quelle del settore privato e, nell'ambito del pubblico impiego, tra amministrazioni centrali ed enti locali. Infine, il Governo, definendo, attraverso il "Documento sulle linee generali e sulle priorità dei rinnovi contrattuali per il quadriennio 2006-2009", la propria strategia negoziale, ha pienamente tenuto conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento al profilo della contrattazione integrativa. PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Scanu e mi complimento con lei anche per la sua capacità di sintesi e di valutazione politica.

mi farebbe piacere dichiararmi soddisfatto, innanzi tutto per onorare la cortesia con la quale mi ha risposto e, in secondo luogo, per il rispetto che debbo alla provvidenza. Purtroppo però, per non essere fariseo, per non essere fariseo, non posso proprio dichiararmi soddisfatto. Al più, posso dirle questo: ho molto più apprezzato l'intervento a braccio, nel quale ho trovato schiettezza, anche se non sempre elementi di condivisione, che il trattato di cui successivamente ci ha voluto dare lettura. Vista la sua cortesia, mi dispiace di questo rapporto univoco che lei ha evidenziato all'inizio. Resta il fatto che attraverso una sfida io avrei voluto farlo diventare bilaterale e lei invece, rifiutandosi, insiste perché rimanga univoco. Penso che la politica non sia una scienza esatta, ma la matematica sì. Le ho presentato dei dati (non degli *slogan* demagogici) che non sono stati contraddetti, semmai letti sotto un'altra ottica, cercando invece di far passare la matematica come una scienza inesatta. Da quei dati emerge che il pubblico impiego è una categoria protetta. Non so se ve ne siete accorti, al Governo, ma non siamo solo noi dell'opposizione a dirlo. La stessa affermazione, utilizzando piuttosto che le parole un altro mezzo di espressione sonora, il fischio, ve l'hanno fatta qualche mese fa a Mirafiori e ve la ribadiranno, in maniera ancora se verranno resi noti i dati che riguardano gli aumenti salariali nel pubblico e nel privato. Lei ha parlato di un'azione di rilancio della pubblica amministrazione. Io ritengo che questa azione avrebbe necessitato mettere sui due piatti della bilancia da una parte dei possibili aumenti salariali e, dall'altra, una discussione seria sull'ammodernamento e sui cambiamenti da apportare nella pubblica amministrazione, affinché una minoranza esigua non diventi invece l'immagine di un'intera categoria e affinché non diventi senso comune quello che i commentatori della vostra parte politica, non della nostra, affermano: cioè che ci troviamo al cospetto di una pubblica amministrazione composta da fannulloni. Questa è un'ingiustizia, ed è un ingiustizia che avreste dovuto smentire attraverso un atteggiamento differente, mettendo in moto le riforme interne alla pubblica amministrazione, necessarie affinché questa acquisizione di dominio pubblico fosse palesemente sconfitta. In molti ambiti, dalla mobilità alla situazione dei dirigenti, non avete fatto questo: non avete avuto la possibilità, se non la volontà, di fare questo.

entrambe le parti in causa e che non ci sia una predominanza eccessiva di una delle due parti. Capisco che in altro ambito, in ambito completamente diverso (quello del diritto familiare), avete previsto che un contratto possa scaturire anche da una semplice raccomandata inviata da una sola delle parti;

ricevere da parte del sindacato una raccomandata per mettere in moto una unione di fatto. Perché guardi, signor Sottosegretario, di unioni di fatto si tratta. Non dubito del valore scientifico e anche della preparazione di molte delle persone che oggi fanno parte dell'ARAN, ad alcune delle quali sono legato da rapporti personali di lunga data. del discorso è diverso. Lei mi può motivare l'assenza di contrarietà giuridiche, ma non può soddisfare un'esigenza di opportunità politica: non mi può dire che chi fa parte del comitato di direzione o del comitato scientifico di una rivista collegata alla CGIL non ha rapporti col sindacato perché quella rivista viene fatta da da una casa editrice che non è la CGIL. Questo significa ricadere nel fariseismo di cui sopra; e so perfettamente che lei non lo vuol fare. Così come non mi può dire - perché sa perfettamente che la potrei smentire - che sono state cause tecniche quelle che hanno impedito la pubblicazione del rapporto

che a presiedere questa seduta fosse il senatore Baccini), perché nell'ultima parte della scorsa legislatura le assicuro che invece i rapporti trimestrali arrivavano in tempo e forniti di ogni dato per comparto; bastava andare sul sito dell'ARAN per vederli. Faccia una capatina oggi a quel sito: lei vedrà un buco nero, uno di quei buchi neri che la Corte dei conti attribuisce alla a voi tanto cara contrattazione integrativa. Due cose per finire, sempre per la schiettezza del rapporto che si è instaurato: lei conosce molto bene la differenza tra un parere vincolante e un parere consultivo, ma soprattutto conosce molto bene la politica e sa perfettamente quale era la cifra politica della Conferenza Stato-Regioni alla fine della scora legislatura. Non mi venga a dire che c'era un Governo differente, perché ciò vuol dire far torto alla mia intelligenza e a quel rapporto di schiettezza che vorrei si possa instaurare

Ritengo solamente che, a volte, dando magari voce molto onestamente alla sua coscienza, prenda degli impegni, anche nelle Aule parlamentari, e dunque documentabili, che poi non può rispettare.

interrogazioni, do comunicazione all'Aula dei risultati della Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza dei Capigruppo riunitasi questo pomeriggio ha approvato modifiche e integrazioni al calendario della prossima settimana e il nuovo calendario dei lavori fino al 3 maggio prossimo. Nella seduta pomeridiana di martedì 17 aprile si svolgerà un'informativa del Governo sulle vicende connesse alla liberazione del giornalista Daniele Mastrogiacomo. Nel successivo dibattito - che non prevede votazioni - potranno intervenire i Gruppi per 10 minuti ciascuno (15 minuti al Gruppo Misto). Nella stessa seduta potrà proseguire la discussione delle mozioni sull'industria agroalimentare - avviata questa mattina e iniziare la trattazione delle mozioni sulla medicina di genere e sul papilloma virus. L'esame del decreto-legge sul ripiano dei disavanzi nel settore sanitario inizierà nella seduta antimeridiana di mercoledì 18 aprile, aprile, con prosieguo nella seduta pomeridiana e, se necessario, in quella antimeridiana di giovedì 19. Quest'ultima seduta - in relazione ai Congressi di partito convocati - non proseguirà oltre le ore 12. Il calendario prevede inoltre - se possibile nel corso della prossima settimana - i disegni di legge recanti delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca e rideterminazione di alcune deleghe legislative. Si ricorda che il sindacato ispettivo della seduta pomeridiana di giovedì 19 aprile sarà dedicato in particolare a materie di competenza del Ministero della giustizia. La settimana successiva alla prossima sarà riservata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea tornerà a riunirsi nelle giornate del 2 e 3 maggio per la discussione del decreto-legge sui consigli giudiziari, per il seguito di argomenti non conclusi e per l'esame del disegno di legge recante delega sui diritti televisivi del calcio. **Programma dei

il sistema di teleprenotazione delle Ferrovie dello Stato Sipax plus è stato progettato e realizzato per offrire uno strumento di lavoro più consono alle esigenze che le agenzie di viaggio hanno manifestato, sottolineando esplicitamente la necessità di poter accedere a tutti i servizi innovativi del canale Internet con costo gestionale contenuto. Il sistema prevede una serie di funzionalità che il precedente non contemplava: basti pensare ai prodotti offerti sul sito Internet di Trenitalia o a quelli forniti dal *call center* della stessa, ma anche a forme avanzate di tele prenotazione.

Dopo una prima fase, che ha registrato il passaggio dal vecchio sistema al nuovo, Ferrovie dello Stato è intervenuta sia sul dimensionamento delle dotazioni tecnologiche per la velocizzazione del sistema, sia per il potenziamento e l'aumento della funzionalità di gestione, comprendenti cambi, rimborsi, forme di pagamento ed altro ancora. In un secondo tempo, sono state risolte le criticità emerse a seguito degli incontri con gli operatori delle agenzie di viaggio. Il programma di risoluzione delle anomalie rimaste è in corso di completamento. Secondo la società, poi, il sistema Sipax plus è un sistema affidabile e la conferma sta nel fatto che alla fine del 2006 i risultati di fatturato del settore delle agenzie di viaggio hanno registrato un andamento maggiormente positivo rispetto all'anno precedente, consentendo alle stesse di mantenere la propria quota di mercato incrementata ulteriormente con la disponibilità di prodotti e servizi più innovativi.

Credo che non sia questa la sede per polemizzare sulle vicende Trenitalia; abbiamo avuto occasione e modo per parlarne durante l'esame del bilancio dello Stato, sollevando la questione del grandissimo *deficit* di questa società, società, affrontando alcune anomalie, onorevole Vice Ministro, di questa società ed alcune iniziative disinvolte relative alle sponsorizzazioni (cose che non dovrebbero appartenere ad una società interamente pubblica), come quella, per esempio, di Roma Europa festival.

ha affermato che la situazione è migliorata. Eppure, soltanto pochi giorni fa mi sono giunte segnalazioni di disagi lamentati dall'utenza

un sistemo operativo che si blocca spesso, le cui linee cadono. Ogni volta che si tenta di superare un problema, se ne evidenzia uno nuovo e diverso. L'aggiornamento, rispetto ai problemi vecchi, fa perciò emergere altri problemi continui e nuovi. Ritengo che su questo punto, onorevole Vice Ministro, si giochi la credibilità dell'azienda,

Con l'articolo 3, comma 1, sono state individuate le tratte marittime da finanziare al fine di incentivare il trasferimento modale dalla strada al mare nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione europea, secondo la quale una tratta marittima può essere finanziata in presenza di un itinerario stradale alternativo, che renda perciò comparabili i due percorsi e permetta di calcolare i costi delle due diverse modalità di trasporto. L'esclusione delle rotte tra la Sardegna ed il resto d'Italia aveva trovato una giustificazione e una non perfetta comparazione tra l'itinerario stradale e quello marittimo. Tuttavia, al fine di riscontrare pienamente le esigenze sorte dall'utenza ed anche le sollecitazioni da parte delle rappresentanze politico-istituzionali, soprattutto della Sardegna, in data 26 marzo 2007 il Ministro dei trasporti ha firmato un decreto integrativo al citato decreto del 31 gennaio 2007, inserendo anche le rotte «fra i porti della Sardegna» tra quelle meritevoli di incentivazione.

data tempestivamente risposta ad un'interrogazione urgente, da me presentata insieme al collega Delogu. Premetto che ho ascoltato la sua risposta e mi dico parzialmente soddisfatto dalle parole che ho sentito.

sia da un punto di vista ambientale. Parlo della accessibilità marittima ed aerea (passeggeri e merci) dell'isola; parlo della continuità territoriale della nostra Regione nei confronti della penisola e, conseguentemente, dei mercati europei. Questo è stato un tema che ha caratterizzato da sempre ed è stato uno dei pilastri di tutte le intese pattizie Stato-Regione. È stata una delle battaglie fondamentali condotte in cinquant'anni di autonomismo sardo. Tragicamente, un semplice emendamento nella scorsa finanziaria ha, di fatto, modificato lo Statuto,

sia se si tiene conto della normativa comunitaria, in particolare dell'articolo 158 del Trattato di Amsterdam, che riconosce l'insularità come uno svantaggio strutturale, sia se si tiene conto delle conclusioni della Convenzione di Nizza, che concede la possibilità di adottare misure specifiche per risolvere i persistenti problemi delle zone insulari. In particolare, lo avevamo giudicato un fatto di gravità inaudita proprio considerando la situazione infrastrutturale della Sardegna. Nord e del Centro-Nord dell'isola gravitano, infatti, sui golfi di Olbia e Porto Torres, mentre la maggiore densità insediativa e produttiva

La decisione che apprendo oggi dal Governo in qualche maniera costituisce un primo passo verso l'obiettivo di inserire completamente le rotte per la Sardegna all'interno delle autostrade del mare. È chiaro che si tratta unicamente di un primo passo; ne prendiamo atto e continueremo a insistere affinché le altre rotte vengano inserite nello stesso contesto.